sono stati dichiarati ammissibili emendamenti quali il 53.0.200 sulla *class action* o il 54.0.12 sui servizi pubblici locali e il presidente Morando ci ha spiegato che, pur trattandosi di riforme che sarebbe opportuno affrontare in altra sede, hanno però ricadute sul sistema economico e, quindi, possono essere collocate nel disegno di legge finanziaria. Non c'è nel fascicolo degli emendamenti,

bensì di diritto transitorio, volto a permettere la copertura di sedi notarili vacanti da parte di chi ha superato le singole prove di concorso, ma non ha raggiunto un punteggio complessivo secondo le disposizioni originariamente vigenti. Questi requisiti sono stati poi soppressi durante lo svolgimento del concorso; sicché quelle prove oggi consentirebbero di ricoprire utilmente delle sedi notarili.

negozio, mentre basta andare a piazza del Pantheon dove ci sono 50 venditori abusivi che vendono occhiali firmati finti con 500 poliziotti che passano ogni giorno e nessuno dice niente. Inoltre, si continua a mantenere un'organizzazione come quella sindacale in Italia, che fattura ormai intorno ai 1.700, 1.800 miliardi di vecchie lire,

parliamo di associazioni benefiche, ma di associazioni cha hanno dipendenti che pagano, che producono utili e che reinvestono non si capisce dove. Quindi, vi è un buco nero nella nostra società per cui, a fronte di una parte del Paese che deve pagare, strapagare perché con gli studi di settore deve pagare anche di più per avere la sicurezza di non trovarsi in casa la Guardia di finanza a controllare i conti, vi sono poi organizzazioni che fatturano 2.000 miliardi di vecchie lire e nessuno controlla niente. Queste organizzazioni

tutto. Poiché voi siete per l'equità, la giustizia e quant'altro, mi piacerebbe sapere perché continuate a restare su tale posizione. Se un commercialista giovane fa il 740, deve rilasciare giustamente la fattura e pagare le tasse alla fine dell'anno, se lo fate voi attraverso i sindacati niente di quello che viene fatto deve uscire sui pubblici bilanci. Con questo chiediamo che finalmente in Italia non ci siano imprenditori, persone che fanno economie di serie A e di serie B, ma che le regole siano uguali per tutti. In questo caso in Italia l'uguaglianza non c'è perché vi è l'organizzazione sindacale che fa politica, fa gli scioperi generali contro una parte, fa finta di niente con l'altra che ha

razionale la questione dei lavoratori socialmente utili e, segnatamente, di quelli della città di Palermo. Si tratta di un provvedimento inserito

L'emendamento che ho presentato insieme al collega Ferrara è stato poi firmato da tutti i Gruppi politici presenti in Aula ed abbiamo anche avuto un contatto con il Governo

per comprendere anche quale atteggiamento finale tenere al momento del voto. **Saluto

poter meglio portare a soluzione la questione dei lavoratori socialmente utili, in coordinamento anche con gli impegni che devono essere assunti da parte del Comune di appartenenza, in una logica che rifletta una sorta di patto tra il Governo ed

un momento in cui, pochi giorni fa, il CIPE ha disposto l'esecutività del finanziamento per la prima *tranche* riferita al 2007,

Caro relatore, l'emendamento 69.800 risolverebbe la questione dando certezza a una norma già applicata qualche giorno fa.

come è previsto nel comma precedente) e senza che sia prevista l'iscrizione delle somme al bilancio prima di renderle interamente ed immediatamente impegnabili, è contrario alla legge di contabilità. Per questo motivo credo sia opportuno votare contro un articolo della finanziaria, quale il 69, che è contrario alla legge di contabilità.

Signor Presidente, a margine della riunione dei Ministri finanziari dell'Eurogruppo il ministro dell'economia Padoa-Schioppa proprio ieri ha espresso preoccupazione riguarda ai livelli insoddisfacenti di crescita e di competitività del nostro Paese. La nostra opinione è che, fino a quando il nostro Paese non si caratterizzerà per una crescita omogenea, la crescita stessa e il prodotto interno lordo non potranno raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci prefiggiamo. Sotto questo aspetto, l'emendamento 69.0.4 coglie l'opportunità per creare le condizioni per investire sulle aree industriali del nostro Paese prive dei servizi essenziali come acqua,

perché non c'è nessun credito d'imposta al mondo, non c'è nessuna fiscalizzazione e nessuno sgravio di natura contributiva fiscale che possa attrarre imprese fintanto che queste non troveranno delle politiche di contesto adeguate. È un emendamento, quindi, che si muove

perché parliamo di alcuni territori dell'Italia che sono fuori dall'Obiettivo 1; però, di fatto, hanno ancora problematiche che per una determinazione regionale non vengono inserite. Faccio esempi precisi: mi riferisco al Lazio meridionale, così come alla Basilicata, che dal prossimo gennaio 2008 sarà fuori. Lasceremmo

l'appunto, ai crediti d'imposta. Ora, io chiedo l'attenzione e la cortesia di dare risposta ad interi territori che in questo modo andrebbero a trovarsi completamente fuori. chiedo il voto elettronico.

e contiene già una parte importante di quei territori in difficoltà a cui si riferiva il senatore Tofani. Questo emendamento del senatore Tofani amplia ulteriormente l'area estendendola a territori che mai erano stati considerati per gli aiuti comunitari o di Stato. La finalità è apprezzabile, ma qui si porrebbe un problema di quantificazione, di copertura finanziaria e quant'altro. Per questa ragione, pur apprezzandone la finalità, esprimo parere contrario.

sottoscritto, un po' più di Europa in Italia, un po' più di giustizia sociale in Italia, un po' più di efficienza. Il confronto col resto d'Europa mostra come sia urgente da noi estendere gli istituti di *welfare* ai soggetti interessati dai nuovi processi di flessibilità. Al contempo, non si può ulteriormente ritardare l'introduzione, anche nel nostro Paese, di istituti che subordinino la tutela monetaria della disoccupazione alla partecipazione di programmi di reinserimento nel mondo del lavoro. È importante, infatti, che tali istituti recuperino la loro funzione di ammortizzatori sociali aventi carattere temporaneo, liberandoli dal ruolo improprio di sostegno corrisposto per far fronte a forme permanenti di disoccupazione. Nel disegno di legge finanziaria si è ritenuto di non voler affrontare queste problematiche, se non in riferimento - come vedo - a specifici casi, rimanendo in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali che è presente nel provvedimento del *welfare*. Questa posizione di attesa è motivata dalla poca disponibilità di risorse. Tuttavia, signor Presidente, in un'ottica mirata a reimpostare su base pluriennale gli istituti del *welfare* e a programmare in tal senso l'utilizzo delle risorse, il Gruppo Socialista ritiene non di meno possibile dare avvio ad un primo intervento di modifica della tutela dalla disoccupazione, sfruttando a tal fine i fondi europei non utilizzati. Avendo in mente questo obiettivo, il nostro emendamento è dunque costruito su tre punti qualificanti: subordinare l'accesso agli istituti di tutela dalla disoccupazione alla partecipazione a programmi di reimpiego professionale, come avviene in tutta Europa; estendere gli istituti di tutela dalla disoccupazione ai lavoratori subordinati iscritti alla gestione separata INPS, attenuando così un evidente fattore di discriminazione oggi esistente sul mercato del lavoro; colleghi (cosa non secondaria), utilizzare per la copertura le risorse non utilizzate, a volte sprecate dalle Regioni, del Fondo sociale europeo, rimarcando in tal modo come le misure a favore dell'offerta di lavoro sono a tutti gli effetti assimilabili

direttamente unordine del giorno, se ho ben compreso. Su tale atto di indirizzo, così come sul contenuto dell'emendamento, vi è piena condivisione della maggioranza, poiché si tratta di misure - come ha detto il senatore Barbieri poc'anzi - che innovano profondamente sul tema degli ammortizzatori sociali in una direzione assolutamente giusta, introducendo, per esempio, la partecipazione ai programmi di inserimento al lavoro di formazione e riqualificazione, la stipula del patto di

velocemente percorrendo il suo *iter* e che si riferisce ad un patto concluso fra il Governo e le parti sociali. Pertanto, nel ribadire piena condivisione, ribadisco

che si tiene nella Commissione competente e quindi nell'Aula che potrà consentire il recepimento, non siamo più nella fase di redazione del disegno di legge. Invito semplicemente a riflettere

cosa fondamentale, l'utilizzo dei fondi europei e i programmi di reinserimento al lavoro. Non è sufficiente un invito generico, perché abbiamo trasformato gli emendamenti in un ordine del giorno a patto che il Governo, attraverso la sua attiva presenza

Sulla base di questo confronto si è addivenuti ad un testo, poi ulteriormente corretto ed integrato, che adesso è all'esame dell'Aula.

caro Sottosegretario, che vi siano figli e figliastri: giovani lavoratori precari nella pubblica amministrazione, da un lato, giovani lavoratori precari nel settore privato, dall'altro. Non so se sono stato chiaro e quindi lo ripeto: credo che l'impegno del Governo nell'accogliere questo ordine del giorno debba essere più preciso e vorrei che le parole e gli impegni assunti in Senato fossero più vincolanti. Le proposte che avanziamo, caro Sottosegretario,

per fare in modo che il lavoro flessibile nei suoi aspetti negativi non sia scaricato su qualche milione di giovani lavoratrici e lavoratori. Questo è il senso della nostra proposta

comprendo l'obiezione del senatore Angius quando confronta questa disciplina con quella relativa alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione. Appare invero asimmetrica la soluzione che si profila di un intervento volto a trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato quello di persone che spesso non sono nemmeno precarie; lo saranno in futuro perché le norme ipotizzate fanno

relativa alle persone che hanno cessato un rapporto di collaborazione a progetto.

si fa riferimento soltanto alle attività di formazione promosse e gestite dai centri pubblici per l'impiego, nel momento in cui, invece, dovrebbe essere consentita anche l'attività di altri soggetti, come gli enti bilaterali per la formazione o le stesse agenzie private per il lavoro. Credo che questa disciplina dovrà essere affrontata nell'ambito della discussione del cosiddetto disegno di legge per il *welfare*,

di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in quanto non detengono la professionalizzazione richiesta da questo processo di informatizzazione e dalle nuove tecnologie. Dobbiamo allora porci anche il problema di come professionalizzare i lavoratori ultracinquantenni e di come affrontare una questione sociale che ormai è drammatica.

che in tal senso avevamo presentato l'emendamento 62.3, che è stato bocciato dall'Aula, a dimostrazione di una sensibilità e di un'attenzione che non è presente nel protocollo sul *welfare* in maniera chiara e definita, in particolare per questo segmento di precarietà di grande importanza. Mi permetta, signor Presidente, di aggiungere una considerazione.

per affrontare questi temi. Mi auguro, però, che questo confronto si possa comunque aprire, anche se mi consentirà di avere delle perplessità rispetto al prosieguo proprio per le considerazioni che mi sono permesso di fare.

qualsiasi altra ipotesi è esclusa, non capisco perché non si vuol dare attenzione a quei territori che confinano con queste zone, che anche in altre finanziarie abbiamo fatto in modo di tenerle in considerazione, sia pure nei limiti delle normative europee e del *de minimis*. Stiamo parlando, tra l'altro, di un impegno di spesa molto esiguo,

Il Governo, con la precisazione suggerita dal relatore in merito all'assenza di oneri per la finanza pubblica, esprime parere favorevole sul testo dell'emendamento 70.3 e parere conforme al relatore sui restanti

parere favorevole, è nato da un convincimento generale che in Commissione giustizia è stato raggiunto. che accomuna maggioranza ed opposizione rispetto ad un articolo, il 78, che prevedeva il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato. In parole povere, l'articolo prevedeva che nelle amministrazioni pubbliche non era possibile utilizzare un precedente giudicato

di poter abrogare l'articolo. Il parere favorevole da parte del relatore e del Governo conforta tutti i componenti della Commissione e tutta l'Assemblea. Quindi, si procederà di conseguenza. Anche sulla base di quello che ha detto il senatore Manzione, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 78.1, anche perché sia io che il senatore Casson ed altri componenti

la maggioranza e il Governo hanno sperperato miliardi di euro del tesoretto, dei tesoretti, delle maggiori entrate o del recupero dell'evasione fiscale

richieste e indicate come via maestra da parte degli organismi dell'Unione Europea. Facciamo articoli di questo tipo per contenere e razionalizzare le spese, naturalmente sempre a carico dei soliti ignoti, magari gli enti locali, com'è scritto. Questo articolo Questo articolo è contrario allo spirito della razionalizzazione delle spese e va a colpire le spese ormai minute, senza

brevemente per sottolineare come l'articolo 79-*bis* credo contrasti con il precedente articolo 76, che prevedeva un intervento legislativo in materia di immobili e di servizi gestiti dalla pubblica amministrazione. La legge n. 326 del 2003 aveva stabilito, in modo inequivocabile, la vendita degli alloggi militari occupati da personale con titolo scaduto; ne derivano entrate per 480 milioni di euro. Le leggi di assestamento e rendiconto generale riportano il mancato introito di questi incassi per la non avvenuta vendita. Ad oltre quattro anni da detta approvazione, nulla è stato fatto, anche se, in data 2 marzo 2006, il Ministro della difesa aveva inviato per il visto di legittimità e la successiva registrazione il decreto ministeriale con cui venivano dichiarati alienabili 4.493 alloggi. Poi, improvvisamente, appare questa norma; domandiamo dov'è la certezza del diritto, stante che sarà difficile individuare

ai dipendenti del Ministero della difesa. Il problema diventa il seguente: perché si deve attuare un piano di realizzazione? Risposta: perché non vi sono alloggi sufficienti per le esigenze di servizio che oggi si devono affrontare. Ma, allora, è possibile fare un unico articolo in cui si dice una cosa e l'esatto contrario? Perché diciamo esattamente che altri alloggi debbano essere dismessi, lasciati o ceduti con la prelazione nei confronti di chi oggi li occupa. Chi occupa quegli alloggi? Sono militari in quiescenza, pensionati delle Forze armate, che, se andiamo a vedere, a stretto rigore, oggi occupano abusivamente quegli alloggi, perché secondo il loro disciplinare, una volta terminata la funzione, avrebbero dovuto lasciare tutti le prebende e gli alloggi di servizio che occupavano in funzione della qualifica che rivestivano.

contrari all'alienazione, ma non vogliamo che si parta al contrario, cedendo quei pochi alloggi che la Difesa ha ancora a disposizione, che manchino gli alloggi per i militari in servizio e che magari non si riesca neanche a fare una giusta

dell'Aula per invitare i colleghi ad una decisione che riguarda la loro coscienza ed anche per evitare una palese ingiustizia. 79-*bis* parla della vendita di alloggi dichiarati non più utili dalla Difesa...

certo punto, si dice che gli alloggi dichiarati non più utili dalla Difesa verranno venduti con un diritto di prelazione a coloro che già li occupano. nell'ambito della Difesa, vi sono più di 3.000 alloggi occupati abusivamente da persone *sine titulo* che, per legge, debbono lasciarli. Ciò sinora non è accaduto perché la compiacenza di qualche Gruppo politico, come accade anche in questo articolo, ha sospeso gli sfratti. Pertanto, l'Amministrazione della difesa ha dovuto accettare che queste persone, che nel momento in cui per legge dovevano lasciare questi alloggi per consentire ad altri di disporne sono invece rimaste, violassero la legge; e adesso dovrebbero avere anche il vantaggio di poter acquistare l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Ora, molte volte ho sentito la presidente Finocchiaro, che al momento non è in Aula, e tanti altri amici che ho anche dall'altra parte fare delle affermazioni, che ho apprezzato, relative alla deontologia, alla giustizia, ad evitare che da quest'Aula

Facciamo sì che alla Camera possa essere ripresentato un emendamento che escluda il vantaggio dato agli abusivi

di giustizia, corretta, onesta, nei confronti di tutti coloro che, per colpa degli abusivi, per tanti anni non hanno potuto usufruire di quel diritto

questa finanziaria con la complicità della sua Presidenza brillante. Lei è un Presidente che farebbe la gioia di qualunque Presidente del Consiglio ed io la raccomanderò agli aspiranti che conosco, perché si guadagna sul campo la Presidenza del Senato: le finanziarie con lei volano. Quindi, è possibile che i colleghi non si siano accorti del fatto che, articolo per articolo, noi stiamo votando di tutto e di più, persino una sorta di riforma del diritto civile, di cui abbiamo sentito negli interventi precedenti del senatore Manzione ed altri. La suscettibilità dell'Assemblea si è manifestata solo quando insieme, insieme, centro-destra e centro-sinistra, avevamo proposto la riforma di una norma anticontraffazione dei simboli dei partiti. Il ministro Mastella, che è stato l'alfiere della bocciatura di quella norma, si è anche risentito, chiedendo che gli facessi delle scuse. Colgo l'occasione per accontentarlo e porgergli ora le scuse per qualche espressione poco felice, e lo faccio non retoricamente. Resta però un dato:

di non agganciare alla finanziaria anche la riforma della legge elettorale, perché la prosecuzione del dibattito non avrà maggiore credibilità.

una menzione speciale da parte della Corte dei conti come ente che fa esattamente il contrario di tutti quelli che andrebbero soppressi. Cito un passaggio della Corte dei conti, per far capire all'Aula di cosa stiamo parlando. Esaminando la gestione 2003-2004 dell'ente, la Corte sottolinea come, pur in presenza di uno stato di crisi economico-finanziaria, l'attività istituzionale non solo non abbia subito significative flessioni, ma abbia registrato importanti traguardi e la gestione dell'Istituto meriti di essere sostenuta ed incoraggiata dal Ministero vigilante per salvaguardarne il ruolo di attore nella scena culturale e di organismo tecnico-scientifico di supporto alla comunità nazionale nella politica estera.

da svilupparsi entro sei mesi per verificare se ci sono margini per una ristrutturazione o per altri tipi di modifiche. Fatta questa doverosa precisazione, ribadisco comunque un parere di conformità al parere del relatore.

l'emendamento 82.5 del collega Storace, mi chiedo, però, perché insista nel voler includere nella lista degli enti inutili da abrogare l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze. Il senso del mio emendamento soppressivo è proprio quello di togliere questo Istituto, che rappresenta un'eccellenza nel campo delle politiche degli aiuti allo sviluppo e della cooperazione internazionale, internazionale, da questa lista infame, da questa colonna infame degli enti da abrogare. Vorrei ricordare che l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze è stato fondato nel 1904 - lo ricordo ai senatori eletti all'estero - proprio per assistere professionalmente l'emigrazione italiana nell'America latina e in Africa. in Africa. Nel 1938 é stato potenziato e rammodernato; nel dopoguerra ha scelto come missione quella di assistere i Paesi in via di sviluppo,

di un organo deputato all'implementazione dei progetti attraverso la collaborazione con le varie organizzazioni non governative. Vorrei ricordare che questo Istituto ha un personale di 35 dipendenti, possiede un bilancio annuo di circa 3 milioni di euro e riceve commesse tre volte superiori per l'attuazione di progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo, svolti in collaborazione con l'Unione Europea, con l'ONU, la FAO eil *World Food Program*. allora, perché debba rientrare nella lista degli enti inutili; mi chiedo perché, se il Governo vuole rivedere la missione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, non attenda attenda la prevista riforma della cooperazione internazionale alla luce della quale, semmai, rivedere, ripensare e ricostruire il ruolo di questo Istituto.

al comma 3, riguardava (come è stato ricordato) la soppressione di alcuni enti ritenuti inutili. A parte il fatto che si

però, a pagina 985 del volume del Servizio studi del Senato, che molto opportunamente la Commissione ha espunto da questo elenco la Lega navale italiana. Questo mi fa molto piacere. Chiedo se la tabella resta cogente e quindi se la Lega navale è salva. Vorrei anche capire dal Governo chi ha avuto la brillante idea di mettere la Lega navale

**Il Senato approva.**

perché il finanziamento alla ricerca scientifica e a quella sanitaria debba essere devoluto esclusivamente ad enti, e non alla ricerca, per cui temiamo che sia indirizzato troppo a soggetti magari amici e non alla ricerca stessa; perché, infine, siano stati espunti dai dai potenziali titolari del 5 per mille i Comuni di residenza. Sarebbe quindi opportuno riportare la normativa anche allo spirito originario dell'istituto. Infine,

sulla base dell'iniziativa che i senatori della Costituente socialista hanno portato avanti nel corso del dibattito di questi giorni in relazione all'8 per mille e alla non esenzione dell'ICI per gli immobili di esclusivo uso commerciale della Chiesa cattolica.

alla distribuzione dell'8 per mille. Abbiamo un meccanismo che gode di una sorta di doppia indicizzazione, perché legato al PIL e alla base imponibile, che

è che questo meccanismo improprio di indicizzazione va verificato e l'inoptato dovrebbe, a nostro giudizio, andare nella piena disponibilità dello Stato

di rendersi conto che sarebbe inammissibile sottoporlo a votazione, proprio per il vincolo degli accordi internazionali che la commissione paritetica non può modificare.

il senatore Novi. Presidente, noi dobbiamo interrogarci sul perché questo Governo si è appropriato

noi potevamo intervenire con queste risorse per alleviare tali sofferenze e abbiamo ritenuto di non farlo; ha ritenuto di appropriarsi di 129 milioni di milioni di euro. È stato un comportamento immorale, in quanto lo stesso ministro Tremonti quando stabilì

per motivare sobriamente le ragioni per le quali chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G84.100. Avrei voluto votarlo già quando era un emendamento, era un emendamento, ma ciò mi è stato impedito dal fatto che è stato dichiarato inammissibile proprio mentre presiedeva il senatore Calderoli; siccome è molto difficile opporsi alla sua provvidenziale e dirigistica maniera di guidare i nostri lavori, mi ritrovo adesso a sostenere la medesima questione nella forma di ordine del giorno. A mio parere, questo ordine del giorno non è inammissibile e non lo era nemmeno quando era in forma di emendamento, perché non chiede di ridiscutere i trattati, ma chiede allo Stato italiano di essere molto preciso nell'applicazione di questo testo; materia almeno discutibile. sarebbe stato il caso di verificare quanti lo desiderano: non è sicuramente la maggioranza dal Parlamento, ma una minoranza che ritiene di avere delle ragioni civili da presentare,

in considerazione le opinioni altrui. In ogni caso, la mia opinione è che questa materia sia oggi in una certa sofferenza; lo rivela il fatto che ogni volta che se ne parla c'è una specie di tensione in Aula. Ad esempio,

suppone che preghi in latino - avrà anch'egli le sue tentazioni, una delle quali è d'intervenire a gamba tesa (non si reputi irriverente questa metafora calcistica, perché Benedetto XVI vuole che il Vaticano abbia le sue squadre di calcio) nelle questioni dello Stato italiano. E lo fa perché la situazione internazionale è tale che con la vorticosa crescita dell'Islam e l'impossibilità dello Stato della Città del Vaticano di entrare in Europa

chiedo di aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno G84.100, insieme

d'altra parte due fattispecie diverse, allora utilizzerei il suo favore. In caso contrario, mi asterrò per una ragione di equità

Io ho chiesto al presidente Calderoli se intendesse far discutere tutte e tre le questioni insieme e il presidente Calderoli ha fatto un nuovo annunzio. A questo punto, noi stiamo intervenendo e svolgendo le dichiarazioni di voto

Non c'è dubbio che vi è un collegamento tra l'emendamento Vegas e l'ordine del giorno Montalbano; credo che questo collegamento sia nella visione che si ha del rapporto tra Stato e società. Mi sembra che vi siano due visioni contrapposte in quest'Aula. La prima è una visione sussidiaria, la quale lo Stato interviene laddove non vi sono energie nel privato per assolvere a compiti che perseguono il bene comune. La seconda è una visione prettamente statalista. Le considerazioni che il senatore Montalbano ha avanzato in quest'Aula non devono assolutamente...

per cui sono messi sullo stesso piano dichiarazioni di chi ha redditi altissimi e di chi ha redditi minimi, portando ad uno squilibrio nell'attribuzione della quota dell'8 per mille. Queste sono le ragioni che mi inducono a

del giorno G84.100 con lo spirito che viene indicato nella parte in cui viene preso un impegno nei confronti del Governo. confronti del Governo. Non penserò mai che assumere un'iniziativa come questa significhi assumere un ruolo ghibellino piuttosto che guelfo all'interno di questo Palazzo. Credo che sia doveroso esaminare la funzionalità e la producenza di un provvedimento. Ho ascoltato con grande interesse tanto quello che ha detto il collega Ciccanti quanto quello che ha detto il senatore Quagliariello. Ma noto in questo una preoccupazione che non ritengo corrispondente alle finalità che vengono qui indicate, che non sono di stravolgimento dei rapporti,

confessioni religiose ad assumere le iniziative necessarie volte alla modifica di criteri di ripartizione del gettito al fine di stabilire che, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale, umanitario, a diretta gestione statale». Non vedo perché il nostro Stato, che avrà tanti difetti ma almeno doveva avere il pregio di poter interessarsi delle questioni di carattere sociale e morale, rivolte cioè al sostegno di situazioni che possono non essere state previste, non possa svolgere questa attività. In questo caso non è di supplenza, ma di attività diretta. Credo allora di aver fatto puramente e semplicemente il mio dovere. Poiché non ho l'abitudine, non ho l'abitudine, a differenza di altri, di subordinare il mio voto alle firme che esprimo: se firmo un emendamento tengo fede ad esso. Non ho questa visione pendolare della funzione parlamentare. Perciò confermo questo con un certo dispiacere mio di non essere d'accordo con la maggior parte dei miei colleghi. Ma questo mi succede qualche volta ed è un presupposto dei liberali quello di avere qualche volta un'opinione che non coincide del tutto con quella degli altri.

Grazie.

e chiedere, se possibile, l'appoggio per la votazione elettronica. So bene che molte colleghe e colleghi non condividono l'opinione che abbiamo espresso nell'ordine del giorno e so anche d'altra parte che i rapporti tra Stato e Chiesa oggi soffrono di una fase di difficoltà, a mio giudizio per una pretesa ingerenza della Chiesa cattolica nell'azione della sfera e delle istituzioni pubbliche, ma questa è una mia personale opinione che può essere ovviamente non condivisa da molti colleghi. Qui stiamo parlando di una questione molto semplice, rispetto alla quale la discussione tra clericali, anticlericali, credenti o non credenti non c'entra niente. Stiamo parlando di una questione che riguarda l'uso delle risorse, dei denari dei contribuenti italiani, punto. Cioè, stiamo parlando di una questione di soldi di soldi e di una questione di libertà. Noi che cosa chiediamo? Che il Governo, badate bene, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e degli accordi fatti con la Santa Sede e di tutte le procedure garantiste

al fine di garantire che, nel caso di scelte non espresse dai contribuenti italiani, si presume volutamente e coscientemente, coscientemente, queste relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale di carattere umanitario a diretta gestione statale. A me, per esempio, piacerebbe che queste risorse venissero spese per fare case popolari; qualcun altro potrebbe preferire qualche altra destinazione, benissimo.

il quale non può dire che siamo viziati da una sorta di statalismo. Chi vi parla, care colleghe e colleghi, è convinto che lo Stato italiano debba finanziare l'attività della Chiesa, per le sue finalità sociali e per la sua missione di fede. Non so come lo dobbiamo dire in termini più chiari. Sono però anche convinto che lo Stato italiano debba preservare la libertà dei contribuenti italiani. La questione allora non è, come dicevo prima, di lotta di lotta all'ultimo sangue tra credenti o non credenti, laicisti o antilaicisti; parliamo di soldi, dell'uso delle risorse dei cittadini italiani: discutiamo di queste risorse. Voglio segnalare, infine, che la Chiesa valdese, tanto per fare un esempio, non accetta questa ripartizione che viene prevista dalle norme vigenti e infatti usa soltanto le risorse che direttamente i contribuenti italiani le versano deliberatamente e scientemente. Per queste di votare a favore di questo ordine del giorno, per affidare al Governo la possibilità e la facoltà di operare nella direzione che abbiamo detto ed auspicato.

si è rimesso all'Aula, mentre il Governo ha precisato che è disposto ad accettarlo come raccomandazione. Presidente, a questo punto, le chiedo formalmente che si voti anche tale per evitare di obbligare il Governo, anche solo con una raccomandazione, ad un comportamento che magari non rispecchia la volontà dell'Aula. Per quanto riguarda noi, non la rispecchia: noi siamo per un parere contrario a questo ordine del giorno,

vanno bene per tutti, si rispettano e parla un oratore per Gruppo. In questo caso vi sono ancora dei Gruppi per i quali nessuno è intervenuto: si tratta del Gruppo dei

non è assolutamente punitivo: si tratta di una norma di chiarezza in riferimento a chi vuole dare effettivamente ad un credo, ad una fede religiosa, un dato contributo e a chi invece non sente tale questione.

questo tipo di proposte hanno delle ragioni forti nella fede e tra i credenti, perché la comunità cristiana e tutte le altre comunità chiedono innanzi tutto tutto a chi ha fede di credere nello spirito e di contribuire alle necessità della comunità ecclesiastica. Il fatto che la Chiesa cattolica non creda più nello spirito e chieda allo Stato di

del costume e delle credenze del nostro popolo, altre volte invece si parla di ciò che uno Stato autonomo fa con un altro Stato. Questa cosa comincia a diventare intollerabile ed intollerante. Terza questione: io credo molto nello nello spirito che si evolve, credo molto che chi ha la fede avrà la possibilità di far fiorire tutto ciò che la contraddizione della Croce porta (non parlerò mai più di religione, giuro, perché sono contrarissimo); ma credo anche molto che sia un gravissimo errore errore chiedere agli Stati (siamo in piena teocrazia, siamo in Arabia Saudita) che ciò che è credenza diventi legge e, a questo punto, istituzione. Non è solo un'offesa alla laicità dello Stato, è anche un'offesa allo spirito e ai veri credenti. Grazie.

dal *non expedit* risorgimentale siamo arrivati al 1929 prima di instaurare, o meglio ricucire, rapporti diretti tra il mondo cattolico e lo Stato italiano. fare un'analisi, lo Stato ha sempre aiutato, ha sempre ritornato quel maltolto di cui si era detto, con la confisca dei beni dello Stato pontificio, in varie maniere: fino a non molto tempo addietro vi era ancora il Fondo per il sostentamento del clero;

Non solo la Chiesa cattolica, ma altre confessioni che hanno sottoscritto le intese si avvalgono di questo aiuto statale. Ai cittadini resta ancora la libertà di dire no, di chiedere che sia lo Stato a gestire quel loro piccolo contributo alla solidarietà:

della solidarietà e del servizio. Da sempre in questo la Chiesa cattolica è al primo posto per frequenza di interventi, per qualità, per creatività e per inventiva. Certamente non è l'unica, ringraziando Dio, essendoci anche una grande collaborazione da parte di altre istituzioni.

ma c'è al centro la *vexata quaestio* dei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, anche in capo ad un Protocollo d'intesa del 1984. Considero forti le argomentazioni del senatore Ciccanti ha sottolineato l'esigenza di un confronto tra lo Stato italiano e la Santa Sede, affinché si pervenga ad una revisione della ripartizione dell'8 per mille, posto che i soldi derivanti dal gettito dei contribuenti, senza precisa destinazione, già vengono utilizzati dalla Chiesa cattolica e da altre confessioni religiose per fini sociali e umanitari.

Binetti. Il nostro voto sull'emendamento sarà dunque un voto contrario. Il mio Gruppo lascia invece libertà di coscienza nel voto sull'ordine del giorno G84.100,

colleghi, veramente senza far polemica, gradirei capire per qualche nostro collega cosa vuol dire la coerenza. Prima c'è stata un'interlocuzione con la senatrice Franca Rame che ha dichiarato di essere poco coerente. Adesso vorrei capire cosa voterà qualche altro nostro collega qui presente, perché ho in mano un appello scritto in cui si chiede che testualmente, riguardo alla norma del 5 per mille, divenga stabile nella nostra legislazione che per la copertura non vengano previsti tetti o analoghe riduzioni. Questo appello Adesso invece voterà un articolo - probabilmente votando contro questo emendamento e poi votando presumibilmente a favore dell'articolo - in cui si pone un tetto.

quindi, il Governo apre una procedura con la Santa Sede. Il Governo non può rimettersi all'Aula o accettarlo come raccomandazione: dev'essere chiara la conseguenza. Invito, quindi, il Governo a prendere una posizione chiara in materia.

capisco che su un ordine del giorno accolto dal Governo non si potrebbe fare alcun intervento, ma vorrei far presente all'Assemblea che l'ordine del giorno accolto impegna il Governo a considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia,

«impegna il Governo a: considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia e degli accordi finanziari internazionali, alla riduzione del debito ed alla ripresa socio-economica del Paese (come avviene in altri Paesi); operare per definire criteri di partecipazione societaria delle Regioni al capitale sociale della Banca d'Italia». Questo è il testo ultimo, predisposto dal senatore

«premesso che: con la privatizzazione della Banca d'Italia le riserve auree ed in valuta estera, ammontanti ad oltre 60 miliardi di euro, non sono più ritenute nella disponibilità dello Stato e che lo stesso problema si pone per i diritti di signoraggio che la BCE versa alla Banca d'Italia; le acquisizioni, gli accorpamenti e le fusioni bancarie, avvenute ed in atto, rischiano di configurare anomale posizioni di assoluto dominio». Si tratta di una premessa che, se mi permette, fa a pugni con il dispositivo di impegno. Il Governo, in questo caso, si sta comportando in un modo assolutamente contraddittorio, non solo rispetto a come è esteso l'ordine del giorno ma anche alle dichiarazioni, ai comportamenti che ha tenuto sino adesso e alle dichiarazioni che la Banca d'Italia ha tenuto a fare nelle audizioni in Commissione bilancio.

intervenire sull'ordine dei lavori, ma colgo l'occasione per suggerire al senatore Iannuzzi l'ipotesi che sia stato il suo angelo custode, e non un amico clericale, a guidare la sua mano. PRESIDENTE. Ognuno ha la sua interpretazione, senatore Buttiglione. BUTTIGLIONE. Invece, sull'ordine dei lavori, signor Presidente, vorrei farle osservare che gli ordini del giorno che si accolgono o si respingono da parte del Governo non possono essere oggetto di una trattativa privata e segreta di cui l'Assemblea può essere tenuta all'oscuro. Quindi, prima che si decida, tutti i senatori devono essere messi al corrente del contenuto dell'ordine del giorno.

tesa a comprendere come mai la Lega navale, che conta decine di migliaia di soci ed è un vanto per la marineria e il diportismo italiano, fosse stata considerata un ente inutile. Ho chiesto al Governo di dichiararci quale fosse la *ratio* per la quale era stato introdotto questo ente benemerito tra quelli che loro consideravano inutili. Il Governo non mi risponde. Ho lasciato che passasse un po' di tempo, affinché si potesse documentare. Vorrei ora capire se si è documentato. Noi già siamo qui a votare mentre il ministro Padoa-Schioppa non è venuto a dispensarci i suoi soliti sorrisi: dovrebbe essere lui il titolare di questo importante provvedimento, ma non si vede.

la riformulazione di questo ordine del giorno. Non so se sia pervenuta a tutti i Gruppi, ma credo non sia possibile trattare un ordine del giorno così drammaticamente differente dall'emendamento

rispetto alla problematica che abbiamo discusso in Commissione sul divieto di ricorso alla procedura arbitrale per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, pur

per suggerire una correzione al testo dell'articolo 86. Poiché al comma 2 si fa riferimento, a proposito del divieto

"partecipate", il termine "maggioritariamente", perché è evidente che per le società minoritariamente partecipate la norma sarebbe sostanzialmente inefficace. Propongo formalmente questa correzione del testo. partecipate maggioritariamente

affrontando un articolo straordinariamente importante ed originale. Dobbiamo alla fervida fantasia creatrice del ministro Di Pietro se per la prima volta, dal 1865, con l'articolo 86 viene espunto l'istituto dell'arbitrato nelle controversie tra società, imprese e pubbliche amministrazioni. Ove passasse l'articolo 86 e venisse respinta la nostra proposta di soppressione il ministro Di Pietro immagina che, non potendo più far ricorso agli arbitrati, sia la giustizia ordinaria a dirimere le controversie. Nelle condizioni in cui versano i tribunali ordinari del nostro Paese, le nostre corti d'appello, lascio immaginare a quest'Aula cosa accadrà in Italia.

Non ho capito

Presidente, dopo le parole del relatore Legnini, che ha apprezzato l'iniziativa, insistiamo affinché l'Aula possa prendere contezza di un problema. un problema. La proposta emendativa che abbiamo presentato non stralcia il divieto di arbitrato ma tende a non privare le parti di uno strumento agile di risoluzione delle controversie, che si è rivelato negativo quando è stato lasciato alle autonome decisioni delle parti, ma che, incardinato in un'istituzione come la camera arbitrale, può essere di ausilio per il mondo produttivo e soprattutto per le amministrazioni. Inoltre, si riducono i costi di aggravamento degli esborsi delle amministrazioni, prevedendo che restino accollati alle parti gli onorari e le spese dei collegi arbitrali e degli avvocati, diminuendo così l'onere a carico dei bilanci pubblici nel caso di soccombenza

qualche lucetta che fa sospettare che possa esservi un voto dissenziente rispetto al Gruppo, all'interno della maggioranza; inoltre che ci siano dei cori indegni che potrebbero apparire di intimidazione verso chi avesse solo la tentazione di votare in modo

Presidente, l'emendamento 87.3 dispone in una materia che probabilmente è di legislazione esclusiva delle Regioni a Statuto speciale;

decreto Bersani dello scorso anno, la norma cioè che riconduceva entro limiti ristretti l'operatività delle società pubbliche, in particolare, di quelle costituite dagli enti locali. A mio parere, questo problema si pone. Tuttavia, anche in questo caso, considerando che tra poco discuteremo della riforma dei servizi pubblici locali e che questo articolo sarà sicuramente oggetto di diversi interventi di

al parere del Governo;

inammissibile un ordine del giorno che smentisce il Parlamento invitando il Governo a disattendere quanto il Parlamento stesso ha stabilito. Si tratta di un precedente pericolosissimo e credo

questione ipocrita. Ricordo che nella scorsa legislatura, quando la cosiddetta legge mancia si applicava solamente alle opere pubbliche,

perché, se da un lato c'è molto bisogno di opere pubbliche, il criterio di scelta non può essere poco trasparente, ai limiti della mancata trasparenza, come è stata fino ad oggi purtroppo l'assegnazione di questi fondi, avvenuta avvenuta con il meccanismo della cosiddetta legge mancia. Quindi, pur riconoscendo l'utilità di molti interventi, abbiamo sempre contestato un metodo che non si basava su criteri di urgenza e di selezione, mettendo a confronto tutte le esigenze dei nostri territori, ma semplicemente di chi stava seduto in quella Commissione. In tal senso condividiamo l'iniziativa del Gruppo dell'Italia dei Valori e la sosterremo pienamente. Presidente, ci dichiariamo favorevoli alla riformulazione proposta dal relatore, impegnando il Governo ad assumere iniziative per riformulare e rivedere la materia in quanto - dovete saperlo tutti - ci sono già dei procedimenti pendenti per appalti e degli impegni

Non vi rendete conto quindi di che cosa significhi cambiare una situazione *in itinere*, in corsa. Sono d'accordo sul fatto che si disponga per il futuro, ma si tenga presente quello che già è stato definito, e mi associo alle parole del

che hanno l'obbligo di eseguire la legge, devono farlo non in base ad una norma di legge, ma ad un ondivago capriccio di un ordine del giorno. Vorrebbe dire che si spendono dei soldi senza una base legislativa o per una finalità ancorché nobile diversa?

Presidente, credo che il senatore Vegas abbia tutte le ragioni di questo mondo. Capisco che la Presidenza, dopo aver dichiarato che l'ordine del giorno era ammissibile, ha ora qualche problema

del giorno vi sia un qualcosa di enormemente sconveniente e mi dispiace che ancora nessuno abbia sollevato tale questione, né il relatore, né la Presidenza, tantomeno il Governo. Si parla infatti di «legge mancia»: ma mancia a chi? Mancia a che cosa? Dove sono i camerieri? C'è un Governo che si siede a tavola e qualcuno che lo serve? *(Applausi dal Gruppo FI).*

vi sono Comuni, enti pubblici e associazioni pubbliche che hanno, in forza di decreti regolarmente adottati dal Ministero dell'economia, nascenti da indirizzi parlamentari, impegnato queste somme, anche perché

che fine fa l'eventuale opera, appaltata o meno. Mi rimetto anche alla sensibilità del relatore. Facciamo in modo di evitare di destabilizzare un sistema Italia con un ordine del giorno (che, tra l'altro, è inadeguato a livello di fonti normative per abrogare quella norma),

Presidente, mi scusi, noi siamo stati in Aula tutto il giorno e anche ieri; siamo stati anche abbastanza attenti, ma non c'è nessuno del mio Gruppo che si sia reso conto del fatto che la Presidenza ha fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti. Può darsi che sia colpa nostra, però, gradiremmo capire quando è stato detto questo, perché a noi non risulta. Se invece è così, chiediamo un tempo minimo per poter presentare

Il relatore ha presentato all'articolo 91 un emendamento piuttosto significativo, questo è avvenuto nel corso del pomeriggio. Non ricordo se in quel momento presiedeva il presidente Calderoli o qualcun altro; comunque, é stato presentato questo emendamento.

per venire incontro alle esigenze sue e di quanti fra i colleghi volessero emendare il testo del relatore. Francamente, più di quello che sto facendo non riesco a fare Prendo atto delle sue comunicazioni, ma prendo anche atto del fatto che c'è una richiesta del senatore Tofani di procedere.

Lega Nord. Al fine di evitare ulteriori discussioni e incidenti, prolungo il tempo per la presentazione dei subemendamenti di un'altra ora;

che in ordine a tale questione (che mi appare in larga misura populista, ma rispetto alla quale posso anche consentire a discutere rispetto a una soluzione che mi sembrava garbata, tenendo conto di una serie di posizioni),

dove ho avuto l'occasione di rendere omaggio ad un illustre esponente del mondo sindacale quale fu Giuseppe Di Vittorio. Nel filmato della CGIL che ricordava le vicende di Di Vittorio mi ha mi ha colpito una sua frase che diceva: «La nostra richiesta di avanzamento non deve suonare come un volere la regressione rispetto agli altri». Francamente, in questo caso bisogna rispettare quanto c'è. C'è anche un altro elemento che mi sconcerta. Noi dovremmo (badate bene)

e tra l'altro questo si sposa con le esigenze di trasparenza e di tempo per la presentazione dei subemendamenti cui lei si è riferito, mi sembrava ragionevole e razionale proporre questa soluzione, con

Presidente, vorrei comunque invitare i colleghi ad aprire il fascicolo del disegno di legge e a confrontare la norma originaria con quella uscita dalla Commissione. Siamo davvero giunti ad una furia iconoclasta che vuol colpire in maniera drastica qualsiasi attività pubblica, prevedendo però delle deroghe (quale quella segnalata dal ministro Mastella)

Presidente, chiedo un attimo di attenzione, perché la questione sollevata dal collega Salvi è molto importante, di ordine costituzionale. L'articolo 91 è stato presentato come articolo votato in Commissione.

ha parlato a nome della maggioranza, della Commissione o del Governo? Ora, il ministro Mastella si è espresso in senso contrario. Vorremmo capire se siamo in presenza di un contrasto tra la Commissione e il Governo un problema di minoranze all'interno della maggioranza. Comunque, mi sembra una situazione molto singolare, dal punto di vista costituzionale. Non è solo il ministro Mastella che deve dire se parla a nome del Governo o no; fino a quando il Ministro siede lì, credo che parli a nome del Governo, credo.

Quindi, chiedo che il relatore chiarisca se ha presentato il suo emendamento a nome della maggioranza oppure

Una volta letta la proposta, il Gruppo Alleanza Nazionale non ha bisogno di presentare subemendamenti e quindi non ha neanche bisogno della sospensione di un quarto d'ora che era stata chiesta.

Presidente, nella giornata di oggi più volte anche autorevoli Presidenti di Gruppo dell'opposizione hanno sottolineato come all'interno della maggioranza, a distanza di breve tempo, si manifestassero cambiamenti di opinione; mi consenta di registrare, con simpatia, che questo accade, legittimamente, anche all'interno dell'opposizione,

perché quello che intende fare il Gruppo Alleanza Nazionale ovviamente è nelle mani del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma

in questo mi sembra debba esserci una coerenza nel concedere il tempo necessario per la presentazione dei subemendamenti.

possibile procedere con l'esame degli articoli successivi. Il presidente Matteoli - almeno fino a questo momento ha sostenuto la tesi che non fosse possibile procedere con gli articoli successivi in presenza di un tempo - che prima indicava in mezz'ora - necessario

e si chiede contemporaneamente di non passare all'articolo 92, l'unica soluzione è sospendere i lavori per il tempo necessario

Ovviamente, il mio Gruppo sosterrà le decisioni che la Presidenza vorrà adottare, nel senso che se vengono fissati,

con grande onestà culturale e intellettuale, ha sottoposto all'Aula una sua opinione di merito che non c'entrava nulla con l'accantonamento né con i subemendamenti, ma entrava nell'argomento.

peso all'interno della maggioranza, tant'è che il Presidente della Commissione bilancio è intervenuto per dire che, a maggior ragione e in maniera trasparente, la maggioranza insisteva

Se poi si tiene conto che sono le ore 20 e che la seduta dovrebbe terminare alle ore 21, le due cose potrebbero coincidere

sul suo testo ci possono essere legittimamente opinioni diverse, pur dovendo io precisare, in risposta alle affermazioni del presidente D'Onofrio, che, ovviamente, ho presentato quell'emendamento a nome della maggioranza. Naturalmente, tutte le opinioni sono legittime ed è giusto e utile che vengano approfondite nell'arco di un paio d'ore. La fissazione di questo termine per i subemendamenti, che costituisce una sua precisa prerogativa, farebbe superare anche il problema dell'accantonamento.

e ho capito anche qual è la posizione della Commissione. Non ho capito qual è la posizione del Governo. Voglio riprendere ciò che ha già detto il senatore Castelli: il Governo si deve esprimere, deve dirci se la posizione dell'Esecutivo è quella del senatore Mastella o quella del relatore o è una terza altra ancora. Noi abbiamo bisogno di sapere cosa pensa il Governo. Capisco che la mia domanda può essere in qualche modo assorbita da questo non inedito ostruzionismo della maggioranza che, non sapendo cosa pensa, cerca di guadagnare tempo per vedere se riesce a venire fuori dalla trappola nella quale essa stessa si è cacciata. Tuttavia, per un regolare andamento dei lavori, abbiamo che il Governo si esprima. Non so chi sia in questo momento il Governo in quest'Aula.

una decisione comune. Abbiamo svolto una discussione sull'ordine dei lavori, soltanto un collega nel merito, il senatore Mastella, ha espresso un parere sull'articolo 91.

l'emendamento 91.850, non meno rilevante dell'articolo medesimo, rispetto al quale la Presidenza aveva concesso un certo termine per la presentazione di subemendamenti.

Al fine di consentire ad altri Gruppi di poter presentare altri subemendamenti, la Presidenza aveva proposto, su sollecitazione del relatore, l'accantonamento dell'articolo 91. l'accantonamento dell'articolo 91. Su tale accantonamento, diversi Gruppi dell'Aula si sono sostanzialmente dichiarati contrari.

qualora l'accantonamento dell'articolo 91, che è stato proposto dal relatore e sul quale si è dichiarato favorevole il Governo, venisse accolto, la proposta della Presidenza è quella di chiudere la seduta, al fine di consentire, sino alle ore 20,30‑20,45, ai Gruppi che intendano farlo, di presentare subemendamenti,